Grazie.

per impedire che consiglieri di una società controllata si trovino anche nel Consiglio di amministrazione della controllante. Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, occorre premettere che, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prevede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse. La verifica dei citati requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari; infatti, spetta al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di sorveglianza o al Consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia degli intermediari, interviene la Banca d'Italia pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti. Analoghe modalità sono previste per la sospensione temporanea della carica, ai sensi del citato articolo 26 del Testo unico bancario e dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale n. 161, in caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal predetto articolo 5, ovvero nel caso di applicazione di misure cautelari di tipo personale. In proposito, giova segnalare che il Governatore della Banca d'Italia, nelle considerazioni finali espresse nel maggio 2010, ha dichiarato che la normativa sui requisiti degli esponenti aziendali è un fondamentale presidio della sana e prudente gestione degli intermediari e una garanzia per la stabilità degli stessi; in tale ottica, ha auspicato l'introduzione nel nostro ordinamento, in linea con quanto previsto in altri Paesi, di un potere di rimozione in capo all'organo di vigilanza dei responsabili di gestioni scorrette o altamente rischiose, prima che la situazione si deteriori gravemente e si debbano perciò attivare provvedimenti di rigore. Con specifico riferimento alla vicenda della Banca popolare di Spoleto, la segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha precisato che la Banca d'Italia, in esito agli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti nel 2010, ha chiesto all'intermediario in questione di adottare un articolato piano di interventi che preveda, tra l'altro, un significativo ricambio nella composizione dell'organo amministrativo, a partire dai componenti di vertice dello stesso. In data 15 febbraio 2011, il Presidente e il Vice presidente vicario del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Spoleto hanno rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi e il primo anche dalla carica di consigliere di amministrazione. La Banca d'Italia, inoltre, ha avviato, nei confronti degli esponenti aziendali della banca in questione, la procedura sanzionatoria amministrativa per le carenze emerse nel corso dei citati accertamenti ispettivi.

c'è sempre la presunzione di innocenza, ma la Banca d'Italia ne ha chiesto la rimozione - sfiduciano il Consiglio di amministrazione della controllante, che detiene il 51,22 per cento della Banca popolare di Spoleto, e si insediano in quella posizione. A questo punto nasce il legittimo sospetto che, per interposta persona, continuino a governare la Banca. Banca. È evidente che ci troviamo di fronte a un caso in cui le raccomandazioni dell'organo di vigilanza, nella fattispecie la Banca d'Italia, uno dei più prestigiosi

presentata. Mi riferisco all'interrogazione del senatore Rutelli in merito alla nomina del direttore della Fondazione Aquileia. A tale proposito, preciso che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia ha personalmente incontrato il direttore della Fondazione Aquileia nell'incontro ufficiale in data 24 febbraio 2011 e successivamente in data 18 marzo 2011, sul tema del conferimento alla Fondazione dell'immobile costituito dall'Essiccatoio tabacchi nord destinato a centro visite dell'area archeologica. La discussione svolta in quella sede ed il testo predisposto dal direttore della Fondazione hanno reso possibile la sottoscrizione, tra il direttore regionale ed il presidente della Fondazione, di un atto di intesa nel comune convincimento che l'ex Essiccatoio, attualmente di proprietà demaniale ed assegnato al Ministero per beni e le attività culturali, debba al più presto essere rimesso in pristino per consentirne per consentirne la migliore e più diffusa fruizione da parte dei cittadini, turisti e visitatori. L'atto di intesa esprime inoltre il concorde intento di assegnare l'immobile, che rappresenta un elemento importante nel contesto dello sviluppo e della valorizzazione della città di Aquileia e del suo vasto patrimonio storico, culturale, architettonico ed archeologico, alla Fondazione; con ciò avviando a soluzione un annoso problema seguito con attenzione da questo Ministero che esprime, pertanto, la propria soddisfazione circa la collaborazione intrapresa con la Fondazione Aquileia e particolarmente col suo direttore. Avete capito? Grazie. lei stesso ha constatato. Ovviamente do la parola all'interrogante.

Ci siamo scandalizzati della vicenda di Pompei, e arriviamo a questo. quale riguarda un argomento specifico e particolarmente delicato. Tra l'altro, abbiamo gridato allo scandalo per la vicenda del crollo di Pompei e quindi è stata prestata anche un'attenzione particolare

un certo tipo di titolo, siamo preoccupati e vorremmo chiedere al ministro Galan, che ha preso impegni solenni su queste vicende, un atteggiamento più attento sotto tutti i punti di vista. Se Se il buongiorno si vede da questo pomeriggio, qualche preoccupazione in più l'abbiamo.

volte a conoscere gli eventuali progetti di recupero del teatro Giuseppe Verdi di Terni e se il Ministero per i beni e le attività culturali non ritenga possibile utilizzare i fondi strutturali europei per concorrere al restauro dell'immobile interessato,

tuttavia causato danni gravissimi al pregevole teatro, che venne in gran parte distrutto; del fabbricato del Poletti si è conservato soltanto il prospetto principale. La parte restante del teatro venne ricostruita nel dopoguerra, su progetto di Leoni, senza tenere conto del disegno originale del Poletti. Attualmente il teatro risulta inutilizzato e necessiterebbe di interventi di riparazione, manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza. Il crollo, verificatosi il 15 gennaio scorso, ha interessato una porzione di controsoffitto nel prospetto principale che costituisce la sola parte ancora conservata del fabbricato ottocentesco. Il Comune di Terni, in accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, ha provveduto a far eseguire gli interventi necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità

I primi lavori necessari per la riparazione del teatro Verdi di Terni sono già stati appaltati con un finanziamento di 300.000 euro da parte dell'amministrazione comunale di Terni. La locale Soprintendenza assicura ogni collaborazione al riguardo, ma l'ipotesi di un finanziamento per il restauro del teatro Verdi, a valere sui fondi strutturali, appare di difficile attuazione in quanto questa Amministrazione non è titolare di programmi FESR. Ringrazio il sottosegretario Giro anche per l'esaustività con cui ha trattato il tema. Mi dichiaro parzialmente soddisfatta in merito alla risposta, perché in realtà la mia interrogazione

permetterne la fruibilità a 360 gradi, ma soprattutto far sì che questo teatro possa di nuovo conformarsi alla progettazione dell'architetto pontificio Poletti e che risale al 1840 circa. Proprio in un contesto ed in un periodo in cui purtroppo le Regioni si vedono bloccate nella disponibilità dei fondi FAS, che potrebbero essere orientati anche all'utilizzo in questi particolari casi anche alla valorizzazione del patrimonio esistente, in un periodo in cui il Ministero dei beni culturali si vede sempre più sottrarre funzioni fondamentali e le missioni di spesa sono decurtate, come ha ben stigmatizzato anche il nostro Gruppo parlamentare nelle occasioni in cui è stato reso reso possibile recentemente, sarebbe per noi importante che il Ministero si rendesse conto che comunque si devono mettere a sistema tutte le risorse possibili per poter fare un intervento di questo tipo, così determinante e significativo per la città di Terni. Si parla di circa sei milioni di euro, il Comune ha già stanziato 300.000 euro, come giustamente lei ha detto, la Regione si impegnerà per quanto possibile, i programmi

riscuotere. Onorevole Sottosegretario, anch'io mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta. In verità, fin dal 18 gennaio 2011, cioè nei giorni immediatamente successivi al crollo di parte delle strutture di copertura del teatro

un approccio un po' diverso, anche con qualche punta polemica verso gli enti locali. Infatti, nel momento stesso in cui, in sintonia con la gentile collega, sollecito l'autorità governativa centrale a fare ogni sforzo e a ritagliare ogni spazio

In questo momento ucciderei un uomo semimorto, e non parlo dell'individuo ma dell'istituzione, perché la Giunta comunale di Terni è dimissionaria, travolta dai suoi problemi politici, economici ed organizzativi.

non è solo un capoluogo significativo, ma che sta anche tentando di giocare sulla sponda della cultura una ripresa della propria immagine e delle proprie aspettative rispetto alle crisi industriali non lievi che l'affliggono, si trova a non poter disporre di una decente struttura teatrale, ed è quindi nella necessità di delocalizzare anche quel po' di iniziative culturali, teatrali ed artistiche in luoghi assolutamente inidonei o infelici.

A questo punto, dopo aver evidenziato il problema, ci auguriamo che il Governo non prenda le distanze da tale situazione e mantenga un contatto, attraverso i suoi uffici centrali e periferici, con gli enti locali, quindi con la Regione e con il Comune, affinché il problema non sia archiviato: bisogna assolutamente risolverlo in un modo o nell'altro, cercando di realizzare quelle sinergie

tutto ciò sta anche compromettendo programmi futuri. Vi sono infatti delle istituzioni umbre importanti dal punto di vista culturale che potrebbero investire su Terni: pensate alla rassegna annuale "Umbria Jazz", che da Perugia si irradia sul territorio;

è stata svolta in linea con quanto previsto nella nota n. 0129433 del 18 novembre 2009, del Capo dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione. Tale selezione non è riconducibile ad alcuna procedura di carattere concorsuale ed è sottratta a qualsiasi forma di prassi o di norma di carattere generale. Si tratta, infatti, di atti meramente discrezionali effettuati dalle singole amministrazioni tecniche dello Stato, per individuare, al proprio interno, particolari professionalità per ricoprire specifici incarichi presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero, ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici del Ministero degli affari esteri. Nel caso in questione, si tratta di un posto di esperto in politiche di internazionalizzazione, politica promozionale e politica commerciale internazionale, da individuare all'interno delle professionalità del Ministero dello sviluppo economico. In secondo luogo, in un'ottica di trasparenza, l'individuazione della professionalità in questione è stata inquadrata in una selezione interna indetta dal capo dipartimento impresa ed internazionalizzazione del Ministero In tale dipartimento sono confluite le direzioni generali dell'ex Ministero del commercio internazionale, competenti da sempre in maniera esclusiva per le materie di internazionalizzazione, politica promozionale e politica commerciale internazionale. Tale selezione, mirata proprio a valorizzare la professionalità ritenuta più idonea tra quelle presenti all'interno del Dipartimento, per destinarla alla posizione di esperto, è stata gestita da una commissione composta dal direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, dal direttore generale per la politica commerciale internazionale e da un dirigente del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione. L'elenco dei componenti la Commissione è stato reso pubblico con la stessa nota, già citata, firmata dal capo dipartimento. In tale nota sono stati altresì comunicati a tutti i potenziali interessati gli aspetti relativi alla valutazione dei *curricula* e dei colloqui che la stessa commissione avrebbe effettuato con i singoli candidati. I quattro candidati, tutti funzionari direttivi dell'area III - sebbene inquadrati in diverse posizioni economiche, uno dei quali con un incarico dirigenziale *ex* articolo 19, comma 6, sono stati attentamente valutati alla luce del loro percorso professionale e delle loro conoscenze tecniche sulle specifiche materie richieste. L'esito della valutazione è stato quello di individuare - concordemente da parte della commissione - la candidata selezionata come quella più idonea a ricoprire l'incarico di esperto da collocare fuori ruolo presso l'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi, in base alle sue specifiche conoscenze tecniche ed al suo *curriculum vitae* In conclusione, si ribadisce che la particolare tipologia di selezione adottata è riconducibile, come già detto, ad una potestà discrezionale della singola amministrazione tecnica, chiamata al suo interno ad individuare le professionalità più idonee a ricoprire gli incarichi di esperti, in base al già citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Pertanto la stessa procedura comparativa di selezione, peraltro effettuata in maniera trasparente e lineare, non rientra in alcun tipo di procedura concorsuale disciplinata dalla legge, come confermato anche dal Ministero per la pubblica amministrazione e di conseguenza si esclude ogni ulteriore verifica

rispetto delle norme e delle procedure. La valutazione dei *curricula* ed i successivi colloqui, integrati dalla prova in lingua inglese sono puntualmente riportati nei verbali trasmessi dalla Commissione alla Direzione generale competente - D.G: politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi. Si evidenzia, infine, che, alla luce del tempo trascorso dalla conclusione della procedura in oggetto, la citata direzione sottolinea l'opportunità che il Ministero degli affari esteri completi al più presto l'*iter* di competenza, relativo alla nomina del funzionario selezionato dal Ministero, il cui nominativo, peraltro, è stato comunicato alla predetta amministrazione già lo scorso 14 luglio 2010, con nota del capo di gabinetto. Al riguardo, si fa presente che l'esigenza di giungere entro breve tempo alla definizione dell'incarico di cui trattasi deve essere posta

che sembra aggirare il testo principale dell'atto di sindacato ispettivo in merito all'esito di una selezione, che si concludeva con la determinazione di assegnare il maggior punteggio alla candidata vincitrice che aveva la qualifica più bassa. Non è la prima volta, signora Presidente, che il Governo viene a rispondere in quest'Aula con Vice Ministri o Sottosegretari che, come direbbe qualcuno, non c'azzeccano nulla

ha provveduto a un'infornata di nove Sottosegretari, questi possano venire in quest'Aula a rispondere con risposte più puntuali, anche perché - lo

devo rilevare che l'interrogazione presentata nasceva da una richiesta di chiarimenti inoltrata l'8 luglio 2010, non dal sottoscritto,

Non mi sembra, signor Sottosegretario, signora Presidente, che un concorso ad Abu Dhabi sia un bene culturale da proteggere, cui offrire tutela. tutela. Quindi, signora Presidente, oltre ad esprimere insoddisfazione, il mio auspicio è che in futuro si possano effettuare concorsi con maggior trasparenza che anche le risposte possano mettere al riparo i vincitori dai legittimi sospetti. La ringrazio, signora Presidente, e ringrazio anche il sottosegretario Giro.

Grazie.